legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea del Senato è finalizzato a riconoscere il 12 novembre quale Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità il 27 ottobre scorso ed è stato esaminato e approvato senza modifiche dalla Commissione affari costituzionali del Senato dopo un breve ma intenso dibattito nel quale tutte le parti politiche, pur nella diversità delle posizioni, ne hanno condiviso il valore e il significato profondo. La mattina di mercoledì 12 novembre 2003, come tutti ricorderanno, giunse la tragica notizia del vile attacco terroristico al contingente italiano impegnato nella missione di pace «Antica Babilonia», decisa dal Governo italiano per collaborare alla ricostruzione democratica dell'Iraq, per ristabilire in quell'area di crisi condizioni normali di vita e per permettere l'avvio delle attività di ricostruzione fisica, sociale e istituzionale. ore 8,40 di quella tragica mattina di novembre un camion con quattro tonnellate di tritolo scoppia a Nassiriya: la base Maestrale dei carabinieri è distrutta Libeccio - la seconda base dei carabinieri - viene gravemente danneggiata. Persero la vita 28 persone, tra cui 19 italiani: 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e 2 civili. La tragica scomparsa dei nostri 19 connazionali a Nassiriya fu, come ha ricordato il Presidente della Repubblica, un esempio di mirabile dedizione al senso del dovere e una straordinaria testimonianza di amor patrio. Non posso dimenticare l'intenso ed elevato dibattito che si svolse nell'Aula del Senato il giorno stesso della strage. A quel dibattito anche lei,

a offrire il loro olocausto per portare la pace in un territorio martoriato dalla guerra e cure e assistenze ai più deboli e indifesi. Tutta la Nazione si strinse attorno alle salme dei militari e dei civili uccisi e ai loro familiari, il cui dolore composto impressionò e commosse il Paese. Condividemmo lo sgomento per le giovani vite spezzate da un atto terroristico di inaudita barbarie, soprattutto perché l'attacco era rivolto contro uomini che stavano partecipando a una spedizione umanitaria e di libertà, in soccorso di un popolo ferito e prostrato da anni di guerra e di dittatura, in difesa della pace, della stabilità e della sicurezza. Quegli uomini erano andati laggiù su mandato del Parlamento, per proteggere la popolazione civile, per istruire la polizia locale, per garantire i soccorsi, per realizzare, con fatica e grandi rischi personali, la pace in un Paese lontano. Agimmo insieme ai nostri storici alleati per difendere l'Occidente dal fanatismo e dal terrore, che, con la strage dell'11 settembre del 2001, aveva dichiarato guerra all'intera umanità. Pagammo un prezzo molto alto, ma non fu un sacrificio inutile. Gli italiani capirono subito il significato di quel tragico evento, manifestando nelle forme più diverse, ma con la medesima partecipazione emotiva, una sincera e unanime solidarietà alle Forze armate. Per la prima volta dopo 60 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale un senso autentico di appartenenza nazionale, né arrogante, né retorico, si raccoglieva composto sotto i simboli della Nazione e dello Stato. Si capì subito che quel tragico evento acquisiva nella coscienza collettiva un altissimo significato simbolico. Ciascuno di noi sentì, come mai come mai prima di allora, l'orgoglio di appartenere alla Nazione italiana, a una comunità di uomini liberi legati da un destino comune, a una comunità di donne e di uomini che condividono un prezioso patrimonio di valori fortemente condivisi - di valori primari, potremmo dire -, quali la libertà, la democrazia e la pace: valori senza i quali la vita stessa non merita di essere vissuta, perché perderebbe gran parte della sua bellezza. Libertà, democrazia, pace, sono i valori che hanno attraversato la coscienza dei popoli di ogni tempo. nei giorni in cui si celebra il ventesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. La libertà è stata sempre la più grande aspirazione dell'uomo, al punto che per difenderla si doveva anche essere pronti ad affrontare la morte. Il 12 novembre di sei anni fa nel popolo italiano si consolidò il concetto che la libertà, la democrazia e la pace, conquistate con il sacrificio di tantissime vite umane nella Seconda guerra mondiale, non sono valori dati una volta per sempre; sono valori che richiedono un continuo un continuo impegno collettivo perché possono essere sempre terribilmente minacciati. Uccisi mentre erano intenti ai loro compiti quotidiani, i militari ed i civili morti a Nassiriya sono certamente eroi del dovere, sono eroi di un dovere adempiuto con dedizione ed amore in contesti difficili e pericolosi. Impegnati in missioni a rischio, in drammatici teatri di guerra, lontani migliaia di chilometri dall'Italia, questi giovani, come tutti i militari e i civili che operano nelle missioni internazionali,

e la *chance* di un futuro fatto di libertà, di progresso e di democrazia! Quanti hanno potuto sperimentare l'umanità dei nostri militari: stare sempre dalla parte della popolazione civile, rispettarla nelle sue usanze, nelle sue idee, nei suoi orientamenti morali e religiosi, aiutarla a ritrovare il meglio delle proprie tradizioni, in una cornice ritrovata, e spesso mai prima sperimentata, di libertà! Con il loro impegno quei 19 caduti hanno dimostrato che la vita è una cosa seria e che per essere all'altezza dei compiti ai quali si è chiamati occorre sacrificio ed abnegazione. I loro nomi si aggiungono a quelli di tanti uomini che nel corso degli anni hanno pagato con la vita il loro impegno in difesa della pace. Penso ai caduti delle missioni in Libano, in Somalia, in Congo, nei Balcani, penso ai militari del 186° reggimento paracadutisti Folgore, morti il 17 settembre scorso a seguito di un altro vile attentato che ha colpito due mezzi blindati italiani lungo la strada che conduce all'aeroporto di Kabul. Sono tutti eroi del dovere, come ho detto, ma sono anche martiri perché, come ricorda il significato del termine, hanno dato testimonianza di assoluta fedeltà non solo alle stellette che portavano, ma anche e soprattutto ai principi di umanità che ispiravano la loro azione e la missione: vincere la pace, difendere la Patria in un modo tutto nuovo rispetto al passato, difenderla proteggendo in qualsiasi parte del mondo la civiltà e i suoi valori. Abbiamo il dovere di ricordarli tutti. È per questo che, con convinzione, vi propongo di votare a favore di questo disegno di legge. Lo dobbiamo alla memoria dei nostri caduti. Lo dobbiamo a tutti i nostri militari e civili attualmente impegnati nelle missioni di pace. Lo dobbiamo a quanti con il loro impegno silenzioso testimoniano lealtà e fiducia nelle istituzioni. Lo dobbiamo ai nostri giovani affinché anche da eventi così tragici, dall'esempio di questi uomini, dal loro sacrificio sappiano trovare prezioso insegnamento per la loro vita. Ma lo dobbiamo soprattutto a tutti gli italiani.

Signor Presidente, ha un significato scegliere questa data per istituire la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Lo ha indicato il senatore Vizzini; e io ricordo, come penso tutti voi, il giorno della strage di Nassiriya: l'angoscia dopo la notizia, le immagini,

anche quegli obiettivi nazionali che magari possono essere più difficilmente percepibili come immediatamente necessari. Non vi è dubbio che per molto tempo in Italia, anche a seguito delle vicende della seconda guerra mondiale, così come è stato in Germania, abbiamo avuto un'opinione pubblica che difficilmente accettava un impegno che presupponesse l'utilizzo della forza.

vero che può essere difficile capire perché i nostri giovani possano morire lontani, in quel momento l'intera Nazione si è stretta intorno a quel dolore e ha capito il senso profondo del

Recentemente sono stata alla camera ardente dei paracadutisti della Folgore morti in Afghanistan, e devo dire che è stata un'esperienza umana particolarmente toccante

Nel ripensare alla dignità e alla forza di queste famiglie, al sacrificio dei loro cari, nel ricordare questo orgoglio rispetto a loro ruolo e a quello che stavano compiendo, io penso che noi abbiamo la responsabilità di sentirci all'altezza di tanto senso del dovere

Oggi la sicurezza di un Paese non si identifica più nella difesa e nella tutela dei confini. Non esistono - e speriamo non esisteranno più - attacchi militari tradizionali.

però, che deve combattere queste insidie là dove si trovano, si organizzano, si addestrano e fanno proseliti. Non vi è dubbio che in questo caso si devono sopportare infiniti disagi,

dalla memoria della politica italiana. Vogliamo ripristinare la vera natura del nostro Paese, ossia un Paese solidale,

Lo dico senza infingimenti, e non con un discorso di maniera. È vero che ci sono già altre date che ricordano i nostri caduti, militari e civili. C'è il 4 novembre, c'è la giornata dedicata al terrorismo. L'anno scorso, il 9 maggio, il Presidente della Repubblica ha voluto riunire le famiglie dei caduti, le famiglie di tanti uomini e donne che hanno perso la vita, per esprimere loro il cordoglio della Nazione, e abbiamo presentato anche un libro. Si poteva immaginare che il ricordo dei caduti nelle missioni internazionali fosse già - e lo era - compreso nelle date celebrative già esistenti. Ma credo che, con grande sensibilità, il Parlamento, la Camera e il Senato, abbiano voluto istituire nel giorno del 12 novembre una nuova occasione di memoria di tutti coloro, militari e civili - e ad essi accomuno giornalisti e volontari - che a vario titolo hanno perso la vita in in occasione delle missioni internazionali. Il Parlamento ha voluto istituire questa data speciale per mantenere ogni anno, in una occasione simbolica, quella vicinanza della comunità nazionale che si è espressa in maniera plastica, vistosa, assoluta nell'occasione di quel 12 novembre in cui celebrammo i caduti di Nassiriya. Questa data vuole oggi ricordare tutti coloro che negli anni hanno offerto il sacrificio della loro vita per portare lontano dalla Patria quel desidero di pace, di libertà, di democrazia e di giustizia, di cui le Forze armate, ma anche i civili che con essi hanno operato,

dal maresciallo capo Pio Semproni, dell'Arma dei carabinieri, al primo caporal maggiore Rosario Ponziano, del 4° Reggimento alpini paracadutisti, che hanno perso la vita, rispettivamente, in Eritrea e in Afghanistan. Sono vite di uomini che sapevano di rischiare, che sapevano, svolgendo quella loro missione, di dover mettere in conto anche il sacrificio più grande, quello della vita, per rendere onore all'impegno preso, per portare concretamente nei fatti,

il Parlamento - è un momento di unità e non di divisione - per il segno di solidarietà che anche in questa occasione sa rinnovare e che, ormai da non breve momento, vede miracolosamente, Camera e Senato, deputati e senatori, uniti senza eccezione quando si tratta di manifestare la vicinanza

degli italiani sia assolutamente consapevole che le Forze armate rappresentano un sicuro presidio di libertà, di sicurezza, di democrazia e di difesa delle istituzioni.

di chi ha il dovere, ma anche l'orgoglio e la passione di difendere la nostra libertà, di tenere spesso lontano da casa nostra pericoli maggiori con la loro azione, il merito di rappresentare

alle mogli, alle madri, ai padri, ai fratelli, ai figli, agli amici e ai parenti, va il nostro affetto e il nostro giuramento che non li dimenticheremo, li dimenticheremo, che saranno presenti ogni giorno, ma una volta l'anno in maniera più forte e simbolica, nel cuore della Nazione, nel cuore dello Stato: quello Stato e quella Nazione che essi hanno servito con assoluta dedizione. Vi prego, per una volta, di accogliere questo sentimento, che non è di un Ministro o di un Governo, ma di tutto il Parlamento e di tutta l'Italia.

Presidente, onorevoli colleghi, ho solo tre minuti per cui per forza di cose dovrò andare a passo di carica. Gli emendamenti che propongo provano ad allargare rivolta alle vittime coinvolte nelle missioni all'estero oltre che a coloro che sono stati coinvolti involontariamente in attività correlate ed al personale delle organizzazioni non governative che con dedizione si dedicano ad una attività di sostegno. Si tratta di coloro che sono colpiti dall'uranio impoverito e di coloro che sono vittime inconsapevoli di azioni di guerra.

le stragi mortali, dopo le stragi mortali all'ONU ed alla Croce Rossa, pochi mesi prima della strage di Nassiriya, ci fanno dire che anche questa strage poteva essere evitata solo se si fossero prese delle iniziative efficaci a proteggere i soldati in una condizione difficile, in mezzo alla città, senza protezione. Penso che si debba dire in Aula che il Ministro della difesa ed i comandi militari, che pure sono stati raggiunti da un'iniziativa processuale del tribunale militare, hanno la responsabilità di non aver protetto i soldati a sufficienza. È dolente dirlo, però sento il dovere di farlo anche di fronte alle famiglie perché il sostegno morale alla coralità della presenza dell'Italia nelle missioni di pace non può essere privato anche di questo sottofondo critico, se non altro per evitare nel futuro degli errori di misura che potrebbero essere disastrosi. *relatore*. Non entro nel merito delle considerazioni. Vorrei invitare il senatore Pardi a ritirare gli emendamenti per trasformarli eventualmente in un ordine del giorno, tenendo conto tenendo conto che il disegno di legge è già stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento e noi oggi vorremmo, nella giornata cui si celebra il Sesto anniversario della strage di Nassiriya, dare una approvazione definitiva del provvedimento, cioè un segnale concreto con una legge che entri in vigore. Quindi, prescindendo dal merito, non do ma inviterei ad aiutarci a raggiungere questo obiettivo, ritirando gli emendamenti e raccogliendo quanto detto in ondine del giorno che il Governo potrebbe valutare ed accogliere per poter procedere nella direzione che ci siamo dati.

Signor Presidente, signor Ministro, le sue parole che condividiamo ci esimono dal fare una dichiarazione di voto estremamente articolata e celebrativa. Credo

serve non solo a sottolineare l'importanza del 12 novembre per le ragioni fin qui dette, ma anche per farci comprendere come sia necessario in un Paese come il nostro, che purtroppo

ancorata ad un sistema di valori, di difesa di un patrimonio comune, che è lo Stato e che il ruolo di questo Stato non solo all'interno dei suoi confini ma soprattutto all'esterno degli stessi: che possa dare la possibilità a noi ed alle giovani generazioni di comprendere che, al di là dell'impegno quotidiano e individuale di ciascuno di noi, esiste una dimensione più ampia, che è fatta dalla comunità della quale noi viviamo, che ha dei diritti ma anche dei doveri.

Ne ha facoltà. CAFORIO *(IdV)*. Onorevole Presidente, colleghi, io e tutto il Gruppo dell'Italia dei Valori siamo intimamente persuasi dell'importanza, anzi della necessità, del provvedimento in esame. Comprendiamo pienamente che l'istituzione di una giornata che sia dedicata al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace possa servire a richiamare le radici democratiche e pacifiche della nostra Nazione. Occorre, però, mantenere il ricordo sempre vivo, affinché rappresenti l'ammonimento per gli errori commessi e l'impegno a costruire un mondo migliore, e per evitare che questa e altre giornate commemorative scadano nella banalità del semplice anniversario e si svuotino di significato. È, perciò, auspicabile che venga compiuto uno sforzo ulteriore per realizzare progressivamente una memoria, collettiva e individuale, salda e perpetua, che si differenzi da quel genere di memoria incostante consolidatasi negli ultimi anni sotto il dettato di diverse celebrazioni, che rischiano di divenire riti Il provvedimento in esame deve essere applicato in quest'ottica, con questo presupposto. Potrebbe rivelarsi utile, a tal proposito, avviare al più presto, in tutto il Paese e in tutte le scuole, iniziative volte ad alimentare e a tenere viva la sensibilità verso certe celebrazioni: perché è indubbio che i giovani siano elemento indispensabile nella valorizzazione del sistema identitario e valoriale di un Paese. È vitale, per la nostra società presente e futura, che i giovani scoprano, e poi vi riflettano, il sacrificio di questi uomini. Persone come loro, che scelgono di svolgere un mestiere così speciale perché credono nella loro patria, nei valori che essa vuole rappresentare e che si impegna a esportare. Vorrei che i nostri ragazzi, oltre a seguire le vicende dei partecipanti al «Grande Fratello», ricordino, o conoscano per la prima volta, anche le vicende dei soldati caduti per l'Italia, caduti per i giovani, caduti per ogni uomo della terra e per la democrazia. Vorrei che i nostri ragazzi sappiano che si può vivere anche di questi valori. Vorrei che i nostri ragazzi, tutti i giovani che frequentano le scuole del Paese ad esempio, si sentano più vicini, almeno rispetto a quanto non appaia oggi, a questi uomini. Uomini che sono partiti portandosi dietro le loro storie, l'affetto dei loro cari, uomini pieni di sogni e progetti, che coltivavano in ogni singolo momento trascorso lontano da casa, con coraggio e speranza. Quando uno di loro perde la vita, si spezza anche la vita della sua famiglia. La vita di ciascuno, poi, va avanti, come è giusto che sia, ma il dolore è di tutti. E se il sacrificio di questi uomini resterà sempre nella memoria di ciascuno, se sarà, quindi, apprezzato, e se sarà, infine, condiviso affinché ne sia alleviato il dolore, allora una giornata della memoria come questa avrà avuto il senso che vogliamo attribuirgli. Ma il mio Gruppo, nel rilievo di questo disegno di legge, ripone anche un'altra aspettativa che ci riguarda direttamente, colleghi. Dopo sei anni dalla tragedia di Nassiriya il ricordo e il dolore restano, ma emergono anche il dovere e la responsabilità. E noi, che costituiamo il Parlamento, dobbiamo assumerci tale responsabilità prima di ogni altro. Siamo noi, Parlamento e Governo, che disponiamo dei mezzi necessari a rendere le missioni internazionali, in cui impegniamo i nostri impegniamo i nostri ragazzi, uno strumento valido ed efficace per il raggiungimento della pace, per la costruzione della sicurezza e per lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni più dilaniate dalla guerra e dalla povertà. Liberare da questi mali le terre dove ogni giorno i nostri soldati prestano il loro servizio vuol dire liberare l'intera umanità. Per riuscirci occorre un'adeguata politica di cooperazione e solidarietà internazionale. Riteniamo, quindi, che questa sia un'ulteriore occasione per sollecitare un dibattito prossimo futuro circa la strategia che l'Italia dovrebbe assumere all'interno del modello di difesa europeo. Consci delle capacità e delle professionalità delle nostre Forze armate all'estero, dovremo definire al più presto i termini politici e strategici con cui mandarle in campo. È necessario che, entro la fine dell'anno, il Parlamento discuta sulle missioni internazionali e sull'Afghanistan con il fine di smetterla con la cattiva abitudine di procedere al finanziamento di dette missioni con cadenza trimestrale o quadrimestrale o, come con l'ultimo provvedimento, addirittura bimestrale. Serve una legge di riferimento sulle missioni internazionali che definisca una strategia in armonia con l'Unione europea e con gli altri Paesi alleati, come gli Stati Uniti; una legge che definisca più coerentemente le attività da svolgere nei teatri in cui operano i nostri militari, che devono essere teatri di pace e non di guerra; una legge che assicuri la copertura finanziaria per almeno tre anni e non più solo per qualche mese, di modo che la loro azione possa svolgersi in maggiore sicurezza e tranquillità; una legge grazie alla quale, in giornate come quella che vogliamo istituire, il nostro ricordo non debba essere rivolto a più uomini di quanti commemoriamo fino ad oggi. Peraltro, mi ritengo un po' deluso per non aver incluso quanto contemplato dagli emendamenti illustrati precedentemente dal collega senatore Pardi. Ci teniamo, infatti, a sottolineare ancora che al seguito di queste missioni e di quanti vi sono direttamente coinvolti rischiano e a volte purtroppo perdono la vita anche altri civili e operatori di pace. È gente che dà un proprio contributo, al di fuori della sfera militare ma con altrettanto valore. Pensiamo solo a quanti si recano nei teatri di guerra per informare noi su quanto accade e per documentare l'azione dei nostri uomini laggiù. Annuncio, quindi, signor Presidente, che l'Italia dei Valori, essendo del tutto in linea con il provvedimento in questione, voterà favorevolmente al disegno di legge n. 1840. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, la Lega Nord condivide pienamente il provvedimento, con il quale lo Stato intende proferire riconoscenza verso quanti volontariamente, abbracciando la professione militare e accettando lo schieramento in teatri di alto rischio, hanno pagato la loro vita, con molta generosità, come successe tanti anni fa per altri militari. Riteniamo che questo sia un atto dovuto da parte del Parlamento, anche per il fatto che a decidere l'invio dei nostri militari è proprio il Parlamento, in quelle zone dove occorre proteggere, mantenere e restaurare la pace. che ciò costituirà altresì un grande e permanente ammonimento a tutti noi, ogniqualvolta in futuro decideremo di intraprendere un'operazione militare all'estero, tanto più che in questi giorni nei quali rinnoviamo gli interventi attualmente in corso non si può dimenticare un fatto molto importante, ossia che per conquistare la pace la pace le nostre Forze armate purtroppo vedranno - speriamo il meno possibile - sempre e comunque qualche lutto. Questo ci tocca dirlo con la morte nel cuore. Ancora è fresco in noi il ricordo delle celebrazioni che abbiamo fatto qualche giorno fa per il 4 novembre, ricorrenza con la quale si ricordano i morti di tutte le guerre. Mi viene spontaneo pensare

il ricordo dei nostri morti vivrà esclusivamente con il pensiero dei vivi. Pensiamo che il 12 novembre ci metterà una volta per tutte di fronte alle nostre responsabilità, alle responsabilità anche di questo Parlamento. Come Lega Nord voglio sottolineare e ricordare che noi

si è congiuntamente emanato. Cercavamo infatti di ricordare come, oltre ai fatti successi a Nassiriya, purtroppo precursore dei tempi fu una vicenda che

dell'arco costituzionale e poi perché non dobbiamo dimenticare che purtroppo sono caduti anche civili. La data mi fa pensare inoltre sia molto propizia per un motivo, se volete, meramente tecnico: riteniamo che

la continuità di queste celebrazioni farà sì che i nostri giovani, soprattutto nelle scuole, possano capire l'importanza che deve avere

apparenza, del soldo e della partecipazione alle cose solo perché va di moda. voteremo a favore di un provvedimento che ci sembra un giusto e dovuto segno di riconoscenza ai nostri caduti per la pace.

Sono familiari dei nostri caduti, di Nassirya e anche di altre missioni.

il Partito Democratico voterà a favore di questo disegno di legge, condividendone lo spirito e credendo fermamente nel significato emblematico e pedagogico del suo contenuto.

ma è una giornata in cui l'Italia fa memoria di tutti i caduti nelle missioni all'estero. Ricordiamo gli italiani caduti in Iraq, i paracadutisti della Folgore caduti nel settembre scorso in Afghanistan e, per fermarci agli eventi più noti, i tanti nostri soldati caduti nelle missioni in Somalia, nei Balcani, nel Congo e in Libano. Vogliamo anche ricordare tutti gli italiani che hanno perso la vita per la pace, l'unità e la libertà di altri popoli e che non sono mai esistiti nel ricordo collettivo del nostro Paese. È questa una vocazione antica del nostro popolo che nel corso dei secoli si è puntualmente manifestata. Pensiamo ai nostri piemontesi che vanno a combattere in Crimea e pensiamo al contributo dato alla libertà dei popoli dell'America Latina da Giuseppe Garibaldi, una figura sacra alla patria, la cui memoria, signor Ministro, pur essendo stata recentemente impunemente vilipesa, rimane cara alla comune coscienza del nostro popolo. Il Partito Democratico, del resto, non dimentica che anche l'Italia è stata sostenuta da altri popoli nel suo secolare cammino verso la libertà e la democrazia. Noi crediamo che queste occasioni civili siano assai utili per rinnovare un senso profondo di gratitudine per i tanti sacrifici di vite umane che, anche se dimenticati, sono a fondamento dei traguardi civili che oggi sono patrimonio del nostro Paese. Questi sentimenti non sempre sono presenti e vivi nella società del nostro tempo e questa smemoratezza dilagante devasta le nostre radici e spesso fa dei nostri giovani degli sradicati. Del resto, signor Presidente, un popolo diventa Nazione attraverso due strumenti: le idealità e i princìpi della propria Costituzione e la memoria comune, che sono, signor Presidente, signor Ministro, i valori indisponibili a qualsiasi compromesso. A noi non interessano gli aspetti retorici di questa iniziativa legislativa; il contenuto del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare trova per noi valore proprio in questo significato: rinnovare e alimentare una memoria che rafforzi e consolidi le radici unitarie del nostro Paese, non in una visione nazionalista, ma, al contrario, in un'esaltazione della collaborazione fra le Nazioni e tra i popoli, che fa comprendere, soprattutto alle giovani generazioni, come l'intera umanità in fondo sia una comunità di destino. Il Partito Democratico sente soprattutto il valore educativo di questa idea, il cui senso più profondo sta nella presa di coscienza che noi siamo chiamati dalle nostre responsabilità civili e politiche ad interessarci non solo del nostro territorio, e che la nostra cittadinanza democratica non si ferma ai confini della nostra Nazione o, peggio, della nostra Regione. La ricorrenza che oggi istituiamo conferma e consacra che questa idea forte della convivenza civile non appartiene più a scelte personali, non è più appannaggio di alcune culture politiche, ma è patrimonio culturale e politico dell'intera Nazione. Questo non può non essere motivo di profondo compiacimento per il Partito Democratico, che riconosce in quella idea una delle radici più emblematiche del proprio patrimonio ideale. Signor Presidente, noi noi non dimentichiamo che esprimemmo forte contrarietà alla presenza in Iraq dei nostri soldati, perché ritenevamo che quella guerra non fosse stata decisa dalla comunità internazionale, ma fosse un atto unilaterale e che costituisse perciò un pericoloso precedente per gli equilibri internazionali e la pace nel pianeta. Le successive vicende hanno dimostrato che quella posizione non era infondata. Non dimentichiamo che, nei giorni che precedettero la tragedia di Nassiriya, vi erano stati da parte dei servizi segnali su possibili attentati; ma ciò non appartiene al dibattito odierno. La nostra cultura istituzionale ci ha insegnato che, oltre la dialettica politica, quando il Parlamento assume una decisione, essa è legge dello Stato. E quindi i soldati, dovunque siano andati, sono parte di tutti noi. Essi sono figli della nostra Patria, e le loro vite troncate, i loro familiari e i loro bambini appartengono ai sentimenti più sacri e profondi di ogni cittadino italiano. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, stiamo per approvare una vera e propria legge di iniziativa popolare, e non sembri

ricordasse, in maniera ancora più forte di quanto sin qui non sia avvenuto, il sacrificio di suo padre e di tanti uomini che sono caduti. In questo senso il Parlamento recepisce una richiesta

questo provvedimento viene approvato dopo che perfino organi di informazione che non si occupano prevalentemente di tali temi hanno interpretato questo sentimento profondo della Nazione. Qualche settimana fa, dopo le ultime vittime di Kabul, è stato il quotidiano "Il Sole 24 Ore", che notoriamente si occupa

la più drammatica pagina delle missioni militari, ma è ovvio che questo disegno di legge si rivolge a tutti i 139 caduti. La strage di Nassiriya però rappresentò anche un grande momento di commozione e coesione della nostra Nazione. Ricordiamo che quando quelle salme furono portate all'Altare della Patria fu forse la volta in cui quel monumento è stato davvero l'Altare della Patria, con quella coda di italiani che entravano e uscivano uscivano e l'omaggio delle massime istituzioni. Voglio ricordare anche che i Presidenti della Repubblica che si sono succeduti negli anni, da Cossiga da Ciampi a Napolitano, hanno sempre interpretato, in occasioni tragiche il sentimento della comunità nazionale. Nessuno di noi potrà mai dimenticare la scalinata del Vittoriano piena dei fiori che la gente comune andava a deporre in quel momento di grande coesione, e la compostezza della comunità nazionale, pure di fronte ad un momento di dolore che avrebbe potuto

o quella missione, ma in quelle giornate l'Italia tutta si strinse, dimostrando anche la consapevolezza che per la democrazia e la pace nel mondo una grande Nazione, com'è la nostra, deve accollarsi certi rischi, a volte anche pagando il prezzo di Ricordiamo le parole dell'omelia che in occasione dei funerali dei martiri di Nassiriya pronunciò il cardinal Ruini, con un intervento grandemente

pronunciate da un importante esponente della Chiesa. Ricordiamo anche nell'ultima occasione, i funerali dei caduti di Kabul, le parole di monsignor Pelvi, che

la nostra discussione sulla legge finanziaria. Credo che oggi abbiamo fatto una cosa buona, e mi auguro che i familiari delle vittime e i rappresentanti delle Forze armate che sono stati qui presenti con noi questa mattina

con quella manifestazione che nei giorni di Nassiriya, e in tante altre occasioni, il popolo italiano ha dimostrato, proprio qui a motivi polemici, ma qualcuno ha ricordato talune manifestazioni e momenti in cui non c'era una vera condivisione: ebbene, che oggi nel Parlamento ci sia unanimità su questa legge dimostra che la democrazia sa scegliere i propri rappresentanti, e non devo aggiungere altro. In altre fasi, forse, avremo avuto qualche discussione in più, ma sono gli italiani che hanno consentito a noi rappresentanti di essere questi e non altri, unanimi e non divisi; e anche qualche osservazione che è stata mossa era certamente accoglibile.

dei carabinieri caduto a Nassiriya: «Grazie agli insegnamenti e al sacrificio di mio padre siamo riusciti ad andare avanti, per merito anche della vicinanza del popolo italiano, che ancora oggi non dimentica il sacrificio di eroi che hanno perso la loro vita per i valori fondanti della nostra Repubblica, la pace e la libertà». Desidero dunque ringraziare infine anche i familiari. Mi auguro, signor Ministro, che alcune valutazioni un po' burocratiche di qualche generale che pensa più al suo incarico

che a questi fatti: la legge deve essere anche una legittimazione di questa scelta, che spesso è stata contestata con letture francamente un po' burocratiche dei comportamenti dei singoli. Siamo qui a testimoniare questo sentimento di cordoglio, e mi auguro che il 12 novembre degli anni prossimi nelle scuole si ricordino queste pagine e si discuta liberamente delle missioni di pace e della libertà del mondo, e si parli di tanti fatti che la scuola ignora. La legge non ha oneri, non comporta vacanze, non bloccherà nessuna attività, ma credo che dovrà spingere le istituzioni tutte, gli enti locali e il Parlamento, ma anche le scuole, a parlare di queste cose e a ricordare ai nostri ragazzi che si può sacrificare la vita per la libertà di popoli lontani, perché ogni pezzo di libertà è la nostra libertà. Oggi noi siamo quindi orgogliosi e commossi nell'approvare una legge che ricorda dei martiri, ma che è una legge per la libertà. Colleghi, prima di procedere al voto non voglio sottrarmi ad alcune mie personali, brevissime considerazioni sulla significatività di questa giornata. In effetti oggi è un giorno molto importante per noi italiani. Sei anni fa - il 12 novembre del 2003 - il terrorismo internazionale mieteva vittime tra i nostri militari, uomini di pace in Iraq, seminando terrore. Cadevano 19 nostri uomini. In quell'occasione il Paese si strinse unito e si inchinò dinanzi al sacrificio di quei nostri uomini, e si strinse attorno al dolore dei loro familiari.

Con questo voto il nostro Paese dice chiaramente al mondo intero che non intende dimenticare i propri caduti. Oggi la Repubblica, nella sua massima autorevolezza e istituzionalità, dimostra di sapere e volere onorare, doverosamente, i propri caduti in missioni di pace. Di questo non posso che ringraziare l'intera Aula e tutte le forze politiche che hanno condiviso questo percorso.

Già ieri il collega Morando ha sollevato in via anticipata profili di possibile Morando ha sollevato in via anticipata profili di possibile inammissibilità di uno dei due emendamenti, o di parti degli emendamenti presentati, in relazione alla

che hanno implicazioni di carattere finanziario assolutamente evidenti, seppur di dimensioni non rilevanti. Ormai da alcuni anni

Presidente, io ho chiesto a lei di disporre l'acquisizione della relazione tecnica: non può essere la Commissione a valutare. Ormai sono ripetuti

di un argomento estraneo alla materia che noi abbiamo discusso. La ringrazio, signor Presidente, perché sono certo che le sue decisioni saranno sagge come sempre.

Lei ha detto che il termine per subemendare è fissato a mezzogiorno, e che forse verrà esteso

contengono molte disposizioni, alcune delle quali sono particolarmente consistenti perché introducono surrettiziamente per via parlamentare la proposta del Governo di istituire la Banca del Sud. Noi abbiamo l'esigenza di conoscere i tempi di lavoro per poter proporre eventuali modifiche al testo che i relatori hanno consegnato.

infatti, che la conoscenza della compatibilità complessiva che emerge dalla valutazione della Ragioneria generale ci metterebbe nelle condizioni di subemendare in maniera più o meno efficace. questo vorrei sapere come intendiamo lavorare questa mattina rispetto a queste due novità della maggioranza: credo sarebbe utile per tutti e renderebbe anche più facile la nostra attività.

La Commissione bilancio, che valuterà i profili di copertura e quindi la stessa relazione tecnica, è convocata per le ore 15. Alle ore 15 prenderemo in esame sia gli emendamenti

gli emendamenti del relatore saranno già corredati da relazione tecnica e quindi, quando saranno presi in esame,

Però, a questo punto dei lavori d'Aula, gli emendamenti sono ancora vivi.

la sottoscrizione è efficace, a meno che il collega Baldassarri non dica espressamente che rifiuta il sostegno ad una sua proposta emendativa; lo dica e ne prendiamo atto.

Signor Presidente, anche il Gruppo dell'Italia dei Valori, con il permesso del presidente Baldassarri, sottoscrive l'emendamento 3.0.9

Vogliamo chiedere anche noi l'autorizzazione al presidente Baldassarri a sottoscrivere il suo emendamento 3.0.9 ai fini dell'eventuale sottoscrizione, qualora non siano commutati in ordine del giorno, dei due emendamenti

Poiché l'attuale tassazione media, secondo i dati ufficiali, è del 23 per cento, al primo anno, come già detto ieri, si crea la necessità di una copertura tecnica ragionieristica di circa trecento milioni. Per gli inquilini, l'emendamento, nell'attuale formulazione, prevede una deduzione fino a 5.000 euro.

recependo la prudenza ulteriore che emerge palesemente dal giudizio espresso dal relatore e dal Governo, propongo una riformulazione volta a far sì che al primo anno la deduzione agli inquilini possa essere limitata a 1.000 euro; quindi, al primo anno la copertura tecnica di 2 miliardi di euro di taglio di spesa è a fronte di una spesa per la copertura di minor gettito di circa 500 milioni

un aumento di gettito per l'erario che chiunque facilmente può stimare in circa 2 miliardi di euro. Chiedo quindi al relatore ed al Governo un'ulteriore riflessione su tale riformulazione, ispirata ad ulteriore prudenza per l'avvio di questo meccanismo che porterebbe all'emersione di milioni di affitti in nero ed alla regolarizzazione di un settore che da decenni in Italia è pervaso da larghissima illegalità; ciò salvaguardando i conti pubblici, anzi, dando un ulteriore contributo di maggior gettito sin dal secondo anno. Chiunque può dimostrare che quello della copertura al primo anno è un problema tecnico-ragionieristico dell'anno in cui parte il provvedimento, perché sappiamo fin dall'inizio che tale misura reca un maggiore gettito. Quindi, ferma restando la copertura a 2 miliardi ridotto l'effetto immediato di utilizzo delle risorse a 500 milioni di euro, con una garanzia che va da uno a quattro (perché il taglio di spesa è quattro volte l'effetto tecnico‑ragionieristico che si determina nel primo anno), è la consapevolezza che dal secondo anno in poi il provvedimento porta un consistente maggior gettito, per almeno 2 miliardi di euro. Concludo, signor Presidente, ricordando che ci sono voluti più di dieci anni per far capire a qualcuno da qualche parte che il provvedimento sulle ristrutturazioni edilizie avrebbe prodotto un maggior gettito: l'Italia ha perso dieci anni mantenendo in quel settore tutto il nero che c'era, e che ancora in parte c'è. Quando finalmente è stato approvato quel provvedimento, ci siamo accorti che produceva effettivamente maggior gettito. Siamo di fronte esattamente allo stessa problema tecnico. C'è poi un problema politico:

1.000 euro di deduzione agli inquilini per far partire il meccanismo; quando arriveranno maggiori risorse, come arriveranno, il Governo potrà valutare se incrementare negli anni successivi la deduzione per gli affittuari; ma per com'è formulata tale proposta non c'è nessun problema di copertura e c'è un forte intervento a sostegno della legalità.

Per quanto riguarda le proposte da ultimo avanzate dal senatore Baldassarri, voglio solo confermare ciò che anche sul terreno tecnico il senatore Baldassarri ha sostenuto. Quando discutemmo (l'emendamento allora era di un relatore di maggioranza alla legge finanziaria che si chiamava Morando) di introdurre il provvedimento per il 41 per cento di detrazione per le ristrutturazioni edilizie e l'IVA

Ma già al secondo anno dell'adozione di quella norma, l'IVA per attività di ristrutturazioni edilizie, colleghi, aumentò del 200

Questo argomento vale anche per il trattamento fiscale degli affitti, sia l'affitto percepito, sia l'affitto pagato. Per questa ragione, signor Presidente, sono qui ad invitarla, qualora il relatore recepisca la sollecitazione ulteriore

ragione, signor Presidente,

del tutto positivo, sotto il profilo del funzionamento dell'amministrazione. Detto questo, possiamo accantonare l'emendamento, in modo da valutare l'esatta formulazione, considerando tuttavia che, anche se si trattasse solo di 500 milioni di euro (sono sempre 1.000 miliardi del vecchio conio), rispetto all'economia di questa finanziaria è una cifra molto significativa, e mi domando se sia proprio questa l'azione più urgente, quella di favorire i proprietari di casa (categoria alla quale noi ci inchiniamo, ovviamente), rispetto a molte esigenze che, soprattutto per gli strati più deboli della popolazione, forse potrebbero essere ritenute prioritarie.

*(PD)*. Signor Presidente, stiamo ancora discutendo del problema dei crediti della pubblica amministrazione nei confronti delle piccole e medie imprese. Volevo fare due ulteriori considerazioni rivolte sia al Governo che al relatore.

si trovano spesso costrette a scontare, con una decurtazione del capitale del 20‑30 per cento, a soggetti finanziari terzi. Questo vuol dire che l'impresa ha decurtato il capitale, il soggetto finanziario terzo ha il capitale al 100 per cento e non ha alcuna premura

devono pagare interessi di mora su tributi che non riescono a pagare. Mi sembra veramente il paradosso di questo Paese: le aziende alla fine pagano addirittura gli interessi allo Stato.

Signor Presidente, con questo emendamento tutto il Gruppo del Partito Democratico propone di istituire il credito d'imposta per l'occupazione, dando un sostegno a quei datori di lavoro che incrementano i contratti a tempo indeterminato. È un provvedimento che prevede uno stanziamento di 500 milioni di euro per tre anni, perfettamente coerente con le direttive dell'Unione europea, ed è rivolto soprattutto a quelle aree

Credo che tutti dobbiamo porci il problema che questa finanziaria non dà risposte al Sud, non dà risposte all'occupazione e, come è stato sottolineato da tante colleghe prima di me, non dà risposte alle donne e all'occupazione femminile. 3.0.822, inoltre, premia chi investe nell'occupazione rispettando le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori. Elimina, dunque, ogni tipo di intermediazione. Per questo vi chiediamo di approvarlo.

Vice Ministro, non è vero ciò che lei ha sostenuto, o almeno non è fondato. Lei qui non trova nessuno che sta proponendo di ridurre l'IRAP nell'immediato, determinando così un vuoto nel gettito, in attesa di riduzioni di spesa che si devono ancora realizzare, con il risultato, secondo quanto lei sostiene, che le riduzioni di spesa poi non si realizzano, la riduzione del gettito si ha immediatamente e si allarga il deficit. Se le nostre proposte avessero questo carattere, lei avrebbe ragione di dare sulle stesse una valutazione ed un giudizio negativi. Peccato però che questo meccanismo lei lo attribuisca ad emendamenti che non lo giustificano. Non è così.

introdurre o dal lato della riduzione della spesa o dal lato di una diversa distribuzione del carico fiscale (per esempio, di più sulla rendita e meno sul lavoro) misure che creano uno spazio finanziario. Alla condizione - e solo alla condizione - che quello spazio finanziario si determini, gli emendamenti propongono di usare quelle risorse finanziarie per disporre una riduzione dell'IRAP. Non potete cavarvela nel rapporto con il Parlamento, con l'opposizione e con il Paese sostenendo che state respingendo proposte che allargano il deficit, e di conseguenza allargano il debito e mettono a rischio la finanza pubblica italiana. Non potete, perché non è così!

dal lato della riduzione della capacità dei contratti di coprire il mantenimento del potere di acquisto dei dipendenti pubblici. Tra la spesa per il rinnovo contrattuale e la spesa, di cui si parla negli emendamenti, per lavoro dipendente, lei mi insegna c'è una certa differenza. Qui affronto il tema della riduzione della spesa corrente primaria dal lato della spesa per lavoro dipendente, che nel corso di questi vent'anni, senatore Garavaglia, ha avuto un'evoluzione quasi doppia ogni anno in termini reali rispetto all'andamento del prodotto interno lordo. del prodotto interno lordo. Questo significa che quell'aumento di spesa non deriva dai rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici, ma da altri fattori, noi che un po' ci occupiamo di bilancio conosciamo benissimo e sono soprattutto gli effetti di quelli che vengono chiamati "scivolamenti". Pertanto, numero dei dipendenti e "scivolamenti" determinano un andamento della spesa infinitamente più dinamico di quanto non sarebbe giustificato dall'aumento dell'inflazione e dall'aumento della ricchezza nazionale. introdurre, nell'applicazione della legge Brunetta, che è di questo Governo, un meccanismo di obiettivi di risparmio collegati all'attuazione di quella stessa Man mano che quel risparmio si determina (a marzo si farà la verifica di ogni anno) si ridurrà proporzionalmente l'IRAP, eliminandone dalla base imponibile il costo del lavoro. Voi dite di no, ma non potete dire che lo fate per ragioni finanziarie. Dite di no perché avete un orientamento politico preciso: la politica economica e di bilancio di questo Governo - quella sviluppata nel corso di quest'anno e mezzo e di cui la finanziaria del nulla è figlia diretta - non deve cambiare, perché i problemi si risolveranno da soli. Questa è la linea di politica economica e di bilancio del Governo di centrodestra. Non è vero, quindi, quello che ho sentito sostenere, anche da parte di forze dell'opposizione, e cioè che il dibattito è tutto dentro la maggioranza e l'opposizione non c'entra nulla. È vero il contrario. L'opposizione sta dicendo: nel quadro del mantenimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica volete cambiare disegno alla politica di bilancio del Governo, nel senso di ridurre la spesa corrente primaria al fine di ridurre la pressione fiscale, per per scopi di sviluppo, e di aumentare la spesa in conto capitale, a scopi di infrastrutturazione materiale e immateriale del Paese? Voi state dicendo di no a questa politica economica e di bilancio, che non è una politica irresponsabile sotto il profilo degli equilibri di finanza pubblica. State dicendo di no perché pensate che l'Italia potrà parassitare gli interventi di promozione dello sviluppo messi in atto dai Governi di altri Paesi nostri partners nel contesto europeo. sbagliate: ad un certo punto usciremo dalla crisi camminando ancora più lentamente di quanto non facessimo prima della sua esplosione, a paragone con gli altri Paesi, e la responsabilità per le mancate riforme che voi ancora adesso rifiutate di fare sarà interamente vostra.

al comma 18-*nonies* dell'emendamento 2.3000, non so se si tratti di un refuso, ma credo sia prevista un'esenzione per chi acquista tartufi. È possibile? O c'è la citazione di una legge sbagliata?

risorse tolte alle scuole dell'infanzia paritarie che in molti piccoli Comuni sono le uniche. È a rischio, quindi, il servizio pubblico della scuola dell'infanzia in questi

cui parlano di libertà educativa. Abbiate il coraggio di dare almeno gli stessi soldi che il Governo di centrosinistra ha sempre garantito a queste scuole. Parlate un po' meno nei convegni e rispondete con i fatti. È una vergogna che fate chiudere le scuole materne paritarie. Ditelo chiaramente agli italiani!

Oggi sia il Ministero dell'economia e delle finanze che il *call center* dell'Agenzia delle entrate hanno riconosciuto che è necessario

chiesto il voto elettronico in questo ordine del giorno sono raccolti gli obiettivi dei nostri emendamenti, che purtroppo non hanno trovato accoglimento in quest'Aula. Si tratta di una questione molto semplice e mi pare anche condivisibile. Gradualmente - abbiamo cominciato con il settore pubblico e seguirà quello privato - verrà aumentata, per obbligo europeo, l'età pensionabile delle donne, portandola da 60 a 65 anni. Noi finora, fanalino di coda di tutta l'Europa, non ci siamo mai permessi misure a favore delle donne e per meglio rendere compatibile il posto di lavoro con l'educazione dei figli e la

nel periodo e con uno sconto sull'età pensionabile per ogni figlio, da definire. Per ora sono quattro mesi e le donne in Alto Adige giustamente chiedono che per ogni figlio, con il contributo che versano, siano scalati almeno due anni. Tutto questo si potrebbe rivedere.

Si tratta delle risorse per coprire i contratti per la gestione degli appalti dei servizi di pulizia e di mensa nelle scuole. Le risorse sufficienti solo fino al 31 dicembre. Se non verranno stanziate nuove risorse per il 2010, circa 14.000 addetti a questi servizi perderanno il lavoro, verranno messi in mobilità. Faccio presente che dal 1° ottobre

una riflessione, anche eventualmente una riformulazione, ma non una raccomandazione. In tutta la premessa si parla del lavoro svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle zone terremotate dell'Aquila e di quant'altro essi fanno e profondono in tutto il nostro Paese:

non si possa accogliere l'ordine del giorno così come proposto. Stiamo parlando di un fatto che non può non condividersi. I vigili del fuoco provenienti da tutta Italia che si sono impegnati nel terremoto in Abruzzo non sono stati pagati o, non sono stati pagati *in toto*. Non è materia da ordine del giorno: ci voleva una norma, uno stanziamento per provvedere a questa necessità inderogabile. Gli esponenti del Governo e della maggioranza hanno fatto la fila in Abruzzo per osannare i vigili del fuoco, salvo poi non dare le risorse necessarie per farli lavorare in tranquillità.

a mezzo del vice ministro Vegas, si impegna seriamente ad adottare una misura concreta in questa materia, allora posso anche accettare la riformulazione. A me è sembrato che la riformulazione, così come motivata e supportata dalle parole del vice ministro Vegas voglia appunto costituire un'attenuazione di questo impegno.

Se vi è qualche difficoltà temporanea di cassa si vedrà come fare eventualmente con delle dilazioni, come si usa - diciamo - nelle migliori famiglie. Non credo vi siano problemi sotto questo profilo ad assumere alcun impegno da parte del Governo.

l'editoria, una complessa questione, vitale per circa 100 testate. Non vedo sinceramente perché non si possa accogliere come ordine del giorno

sottovalutare l'impegno attivo del Governo in questa materia. sullo stesso l'attenzione di tutta l'Aula e del Governo, con un po' di calma, di serietà e direi anche di rispetto su tale questione. Stiamo parlando del fenomeno della violenza sulle donne.

pertanto l'attenzione sul tema di tutti i colleghi, e soprattutto di tutte le colleghe, perché credo che un ordine del giorno non fa cadere il Governo e forse potrà servire a esprimere una punta di dignità e anche di autonomia.

nell'emendamento del relatore siano previste risorse aggiuntive per le forze dell'ordine. Non posso non notare come per esempio nell'ordine del giorno G2.116 sia indicata una politica di aumento delle risorse destinate ai contratti

con lo stanziamento di 100 milioni di euro, che hanno peraltro una loro finalizzazione precisa, così come previsto dal testo, cioè di finanziare un finanziare un aspetto del rapporto contrattuale del personale del comparto sicurezza, quella tanto controversa questione che attiene alla specificità delle funzioni, che doveva essere anche in passato finanziata e che non lo è stata, è un conto. Se loro ritengono che queste somme siano sufficienti ad esaurire il tema del comparto sicurezza, allora mi sarei aspettato un parere contrario sull'ordine del giorno; se, viceversa, loro ritengono che ci sia la necessità, tra le priorità di questo nuovo tesoretto del centrodestra, cioè il gettito derivante dallo scudo fiscale,

sulla base di quello che arriverà con lo scudo fiscale, ci sarà un impegno riferito anche al riordino delle carriere e quindi ai contratti. È nota la posizione, in particolare, del mio Gruppo, ma adesso parlo come relatore di maggioranza. È chiaro che sulle cifre non ci fermiamo, per cui rimaniamo sulla sulla raccomandazione. Capisco che il senatore D'Alia voglia farli votare comunque, però credo che non ci sia dubbio sull'impegno. È il primo impegno che questa maggioranza sta prendendo, dimostrandolo a ogni piè sospinto, compreso il prossimo emendamento che voteremo.

non mi è ben chiaro il fatto che nei giorni scorsi il Ministro dell'interno abbia detto che nell'ultimo anno sono state confiscate somme pari ad un miliardo di euro e poi si riduce lo stanziamento per il comparto sicurezza per 900 milioni di euro. Questa politica è così contraddittoria che mi fa mi fa venire il dubbio di essere stato preso in giro nel momento in cui il Ministro dell'interno annunciava queste fandonie sui sequestri effettuati e sulle somme confiscate nell'ultimo anno. Reputo offensiva la proposta del relatore e del Governo

intervengo per rivolgermi al relatore e al Governo. Trovo francamente singolare la richiesta di trasformare questo ordine del giorno in raccomandazione quando di fatto - pregherei il relatore

l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è interamente finanziata e che i lavori si concluderanno entro il 2012. Sappiamo perfettamente che non sarà così e credo che l'accoglimento dell'ordine del giorno sia una minima prova di garanzia rispetto a quanto il Governo asserisce. Non solo rimango quindi convinto della necessità di votare l'ordine del giorno, ma francamente consiglierei al relatore e al Governo di accettare l'ordine del giorno che abbiamo proposto.

Presidente, mi corre l'obbligo di rispondere in particolare perché vengo dalla stessa Regione della senatrice Donaggio. Nell'ordine del giorno si stabilisce un impegno sulla spesa e sul ripristino delle risorse;

di un auspicio, di un interesse comune ad intensificare i controlli sulla strada. Il provvedimento rischia altrimenti di caratterizzarsi esclusivamente per l'inasprimento delle sanzioni quale unico deterrente

Senatore Casson,

come raccomandazione, perché è già grave che siano state sottratte risorse per la difesa del suolo e per l'assetto idrogeologico del nostro territorio è gravissimo che non si vogliano impegnare le poche risorse disponibili in maniera ordinata e secondo le priorità di rischio. rischio. Con quest'ordine del giorno si chiede infatti di rispettare le indicazioni dei piani di assetto idrogeologico

Si chiede altresì di agire anche dal punto di vista normativo perché i centri funzionali presenti nel territorio regionale possano essere meglio coordinati con le strutture centrali del Dipartimento della protezione civile, che va potenziato ulteriormente, al fine di attenuare i fattori

**Il Senato non approva.**

si tratta di capire e valutare l'eventuale riformulazione. Sarebbe però assolutamente opportuno - da un lato - un ordine del giorno preciso che si assuma l'impegno di rifinanziare la legge di settore sulla portualità, la quale dal 2002 di fatto non viene rifinanziata; formale ulteriore impegno, dopo quelli che abbiamo reciprocamente assunto anche nelle passate legislature, rispetto ai dragaggi portuali, che costituiscono davvero l'emergenza rispetto al sistema portuale italiano. Sono porti

ad assicurare ai lavoratori l'indennità di vacanza contrattuale. Quindi, con l'ordine del giorno G2.146 impegniamo il Governo al raddoppio delle risorse per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 per il settore del pubblico impiego. Chiedo la votazione nominale

la raccomandazione è reato oppure no? Il Governo ha bisogno di raccomandazioni per fare il proprio dovere e dare risposte ai cittadini italiani oppure è capace di farlo?

testo: ieri un emendamento, presentato dal Partito Democratico, è stato dichiarato non valido, perché non votato da parte della maggioranza e del Governo.

Presidente, speravo vi fosse una maggiore attenzione a questo ordine del giorno, che vuole aprire uno squarcio sul silenzio che da anni c'è sulla sindrome post-polio. Chi è della mia generazione ricorda ancora di bambini morti di poliomielite. Ci sono le persone sopravvissute, verso le quali c'è assoluta indifferenza rispetto alle patologie della post-polio, riconosciute anche in importanti congressi scientifici nel nostro Paese. Da anni i centri di ricerca, cura e studio di questa malattia sono stati completamente abbandonati. Speravo che la richiesta di una maggiore attenzione rispetto alla cura, alla ricerca, all'informazione della classe medica su questo problema potesse essere accettata dal Governo e mi rammarico molto che questo non sia avvenuto. Circa 70.000 persone

non posso accettare l'accoglimento come raccomandazione per alcuni motivi di fondo. Innanzitutto, questa posizione è in netta contraddizione contraddizione con le affermazioni di alcuni illustri membri del Governo, dal presidente Berlusconi al ministro degli esteri Frattini: in alcuni incontri fatti a livello intergovernativo con i rappresentanti del Governo sloveno costoro si sono impegnati a trovare i fondi per coprire le spese di funzionamento previste dalla legge n. 38 del 2001 per la minoranza nazionale slovena. Per quanto riguarda anche la minoranza italiana in Slovenia, c'è stato un preciso impegno da parte del presidente Fini durante il recente incontro con la rappresentanza parlamentare della Croazia, di cui faceva parte anche il parlamentare della comunità italiana, onorevole Furio Radin. Vorrei ricordare ai rappresentanti del Governo che lo scorso anno abbiamo assistito ad un comportamento uguale a questo,

ha garantito gli stessi contributi alla comunità italiana e, nel recente incontro di Brdo, nel comitato interministeriale ha garantito anche l'assetto di "TV-Capodistria". Non sono un'assertrice della reciprocità, però vorrei ricordare al Governo gli impegni assunti.

Presidente, vorrei fare un appello al Governo a rivedere il suo parere. Questo semplice ordine del giorno impegna il Governo a valutare, ove lo consentano le condizioni di stabilizzazione

l'ordine del giorno G2.172 riguarda la questione del Patto di stabilità degli enti locali; se ne è parlato a lungo. È stato richiesto di sopprimere la parte relativa al superamento delle sanzioni, ma restano fermi due punti fondamentali per me e per il mio Gruppo: quello relativo alla revisione del Patto di stabilità interno, al fine di consentire gli investimenti degli enti locali (mi auguro che questo sia possibile fin dalla discussione alla Camera dei deputati anche questo molto è importante - l'impegno al Governo a restituire integralmente quanto dovuto ai Comuni per il mancato gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Era insostenibile anche per la maggioranza la contraddizione tra il federalismo a parole e il centralismo esasperato nei fatti. Questo è il segno che in qualche modo i nostri argomenti cominciano a fare breccia. Non è certo la soluzione del problema, ma la maggioranza e il Governo stiano tranquilli: non molleremo la presa e continueremo a segnalare che è una questione fondamentale non solo per i Comuni, ma per tutta l'economia italiana.

Sì, Presidente, accolgo la proposta del relatore, segnalando peraltro che la precisazione che richiede, e che accetto,

parliamo di provvedimenti sulla velocizzazione dei processi, non dovrebbe sfuggire all'attenzione un ordine del giorno che chiede appunto di migliorare l'efficienza del sistema giustizia.

Non accetto la raccomandazione, nel momento in cui stiamo leggendo il testo dell'ennesima norma vergogna, che determina un omicidio processuale del nostro sistema per favorire un imputato: nel momento in cui presentate questa vergogna, negate le risorse alla giustizia. Vergogna!

il 12 febbraio 2009, è stata presentata una mozione, a firma trasversale, dalla senatrice Boldi, dalla senatrice Bianconi e dalla sottoscritta,

del Governo è conforme a quello del relatore, tenendo conto che

che, tutto sommato, il Governo consideri la sanità come un *optional* per il Paese o comunque che quell'universalismo selettivo, cui fa riferimento il ministro Sacconi, preveda che qualcuno rimanga fuori dal sistema sanitario nazionale. Noi vogliamo ribadire che l'universalismo è

dal presidente D'Alia questa mattina, c'è un problema piuttosto serio. Chiedo quindi alla Presidenza del Senato di concederci altro tempo per la presentazione dei subemendamenti.

se fosse stata violenta! - «finalizzata alla critica della visione di un'Europa priva di quei valori che l'hanno costruita nei secoli: cristianità, Nazione e popolo. I Radicali sono tra coloro che vorrebbero distruggere questi princìpi e svuotare l'Europa, sia spiritualmente che moralmente. Il loro pensiero rispecchia la deriva che l'Europa di Lisbona sta prendendo, scardinare culture e valori millenari. La sentenza della Corte di Strasburgo sui crocefissi è un esempio di disgregazione dell'identità comune ai popoli europei. Non permetteremo a nessuno di imporre dogmi ultralaicisti in Italia e chi tenterà di rimuovere il crocefisso si troverà di fronte a un muro umano guidato dalla lotta studentesca. Con questa iniziativa lanciamo ufficialmente la campagna per riportare i crocefissi nel nostro Paese». In risposta a questa iniziativa, lancio una campagna straordinaria di iscrizione al Partito radicale transnazionale e informo che da oggi pomeriggio a Chianciano si terrà l'VIII Congresso dei Radicali italiani.

non sa come sfamarsi: è un pensiero che mi tormenta e che non ci può lasciare indifferenti. Propongo ai colleghi un gesto di solidarietà, di certo non mediatico, come un digiuno personale, da attuare prima del 16 novembre, quando presso la sede FAO di Roma si aprirà un dibattito sulla sicurezza alimentare nei Paesi poveri.

su una questione che riguarda, ancora una volta, il sudato risparmio degli italiani. Ci sono stati i fenomeni di Cirio, Parmalat e Lehman Brothers ed è stato quantificato che negli ultimi sette-otto anni un milione di risparmiatori ha perso qualcosa come 50 miliardi di euro: i risparmi sudati, i risparmi dei vecchi, le liquidazioni, il sudore della gente. Ora leggo che sarebbe

intervengo per richiamare la sua attenzione, e credo la solidarietà dell'intero Parlamento, nei riguardi del ministro della gioventù,